***Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie***

un ordinato svolgimento dei nostri lavori. Gli orari già indicativamente fissati per le dichiarazioni di voto e per la chiama slitteranno di conseguenza. La seduta è sospesa.

per alcune questioni sulle quali il Governo ha chiesto di integrare l'emendamento c'è stato un preventivo passaggio in Commissione bilancio per i profili finanziari e in una sede informale delle Commissioni 1a e 5a, con i Capigruppo, per i profili di merito. Questo va detto perché, signora Presidente, le cose sono andate tutte esattamente in quel modo, tranne, come è stato osservato nella Commissione, per una sola questione, relativa in particolare alle quote latte, per le quali una riduzione, pure giusta e riconosciuta,

per mera dimenticanza; è stato giusto da parte dei colleghi dell'opposizione osservarlo, corretto da parte del Governo riconoscerlo. Questa è la prima questione fondamentale.

di questo tipo, di lavorare in tempi e con modi il più possibile adeguati alle nostre possibilità, facendo in modo che la presentazione del maxiemendamento contestualmente corredata da relazione tecnica. Solo questo ci dà i tempi necessari per una puntuale valutazione che, come dirò alla fine

tutte e due le Commissioni, quella presieduta dal presidente Vizzini e, in quest'ultima fase, la nostra, e in particolare i colleghi dell'opposizione, hanno avuto sempre un atteggiamento rivolto alla conclusione del provvedimento, senza mai cedere ad un atteggiamento, pur assolutamente legittimo, di carattere ostruzionistico. Quindi, il maggior tempo a disposizione delle Commissioni è utile soltanto ad un migliore approfondimento del lavoro.

esse sono state chiarite da un successivo intervento del Governo; su altre si è continuato a registrare un dissenso: alcuni

(mi riferisco ad esempio al punto relativo al commissario straordinario per Roma), mentre i colleghi della maggioranza hanno mantenuto un parere favorevole. Questo sulla base di osservazioni tecniche che non devo qui ripetere.

Il dibattito è stato particolarmente approfondito in materia, perché si tratta di un emendamento cifrato per 2.800 milioni di euro, quindi una cifra particolarmente significativa. Al riguardo, però, un'attenta valutazione ci consente di dire che non ci sono effetti finanziari, nemmeno di cassa, perché anche l'acconto è fatto per un periodo infra-annuale. Abbiamo svolto alcune considerazioni di merito, che però non sono parte della mia relazione sull'argomento,

dei Comuni interessati dal terremoto dell'Abruzzo, in particolare il Comune dell'Aquila e pochi altri, per cui si è discusso a lungo se le modifiche che la Ragioneria ha richiesto essere introdotte, e che io, all'esito, chiederò al Governo che siano introdotte fossero - come sostenuto da questi colleghi - tali da

ritenuto che le questioni poste dalla Ragioneria non rendano inefficace l'emendamento, ma lo subordinino ad alcune condizioni di carattere meramente finanziario. Questo è stato il senso del dibattito che si è svolto. Devo dire però che siamo stati favoriti dal fatto - ed ecco il senso dell'auspicio rivolto al Governo, che rinnovo, di consentirci sempre di lavorare con i necessari documenti di carattere finanziario - che

di una norma riguardante il tasso considerato di usura nella concessione di prestiti da parte degli istituti di credito e la specifica finalizzazione della possibilità di BancoPosta di acquistare quote di banche, per limitarla ai fini dell'acquisizione del Mediocredito Centrale, passaggio ritenuto dal Governo necessario per la costituzione della Banca del Mezzogiorno.

il Governo ha posto la fiducia, sia modificato per le parti contenute alle pagine 31 e 32 della relazione tecnica depositata agli atti della Presidenza,

fosse da accogliersi. La maggioranza della Commissione si è espressa nel senso del non accoglimento di questa condizione, sulla base del fatto che è l'unica, come potete vedere, che contiene una modifica di carattere testuale, modifica alla quale non sono annessi effetti onerosi certi, ma solo presumibili. I colleghi dell'opposizione ritenevano che anche questo fosse un segnale di allarme

che correggono esclusivamente e meramente questioni di carattere finanziario, con esclusione della sola prima condizione. Ciò significa che quelle parole rimangono nel testo. Ritengo così di aver riassunto, in termini

è puntuale anche nel riferire delle nostre ulteriori osservazioni critiche, diverse da quelle sostenute dalla maggioranza. Prendo la parola non per correggere, o tentare di correggere, quanto detto dal presidente Azzollini, che è perfettamente corrispondente alla discussione da noi svolta, ma per una ragione precisa, riguardante il riproporsi di un problema che, secondo me, deve essere risolto in termini di sistema. La relazione tecnica all'emendamento del Governo interamente sostitutivo del disegno di legge Io ho avuto in mano, come tutti gli altri colleghi della Commissione bilancio, questa relazione esattamente alle ore 16. Si tratta di 31 pagine di osservazioni tecniche analitiche rilevanti ai fini della nostra decisione, da esaminare in un'ora, comprensiva della discussione delle stesse in Commissione bilancio. Così non si può andare avanti. Il Governo si è impegnato a fare in modo che non accada più, ma temo che sia come certi proponimenti. Mi chiedo se, esattamente in via di fatto, e non in via di diritto, come abbiamo fatto quando con il presidente Pera stabilimmo che in queste circostanze si conferiva il testo alla Commissione bilancio per un esame dei profili di copertura finanziaria, non si dovrebbe stabilire che il testo dell'emendamento o del disegno di legge complessivamente, su cui il Governo mette la fiducia, è accettato come base per il prosieguo dei lavori dalla Presidenza solo se è corredato - come stabilisce il nostro Regolamento - da relazione tecnica. Mentre il nostro Regolamento ammette che qualsiasi altra proposta d'iniziativa parlamentare possa essere non corredata da relazione tecnica, nel caso delle proposte del Governo il Regolamento obbliga alla presentazione della relazione tecnica. Bisogna semplicemente, in via di fatto, signora Presidente, affermare la contestualità della presentazione: intanto l'emendamento viene considerato correttamente presentato dal Governo in quanto ci sia la relazione tecnica che lo accompagna. In questo caso, poi, la cosa la cosa è particolarmente sgradevole perché questo testo, con l'eccezione delle norme relative agli istituti di credito, è esattamente il testo degli emendamenti approvati in Commissione. La Commissione ha terminato i suoi lavori venerdì: per quale ragione il Governo non deve essere in grado di presentare la relazione tecnica il martedì successivo al venerdì in cui è terminato il lavoro? Non c'è una ragione sensata. È per questo che mi permetto di suggerire alla Presidenza del Senato

messo alla base del dibattito sulla fiducia in quanto nello stesso momento sia accompagnato dalla relazione tecnica. Così anche questa storia del ritardo finirà.

Senatore Morando, è senz'altro l'auspicio anche della Presidenza che vi sia contestualità tra presentazione del maxiemendamento e della relazione tecnica bollinata. Invito il rappresentante del Governo, onorevole Giorgetti,

finanze*. Le modifiche si intendono recepite all'interno del testo sulla base delle condizioni poste dalla relazione del presidente Azzollini.

prima poste da parte del presidente Azzollini che sono accolte e integrano il testo su cui il Governo ha posto la fiducia, mi permetto di sottoporre all'Aula le seguenti richieste di coordinamento formale del testo e di rettifica di errori materiali. materiali. Nella parte Allegato, all'articolo 2: al comma 1-*sexies,* lettera b), sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «comma 4»; al comma 1-*septies,* sostituire le parole: «presente articolo», ovunque ricorrano, con le seguenti: «comma 1-*sexies*»;

al secondo periodo sostituire le parole: «del citato articolo», con le seguenti: «dell'articolo» e le parole: «nel presente articolo», con le seguenti: «nei commi 6-*undecies*, 6-*duodecies*, 6-*terdecies* e 6-*quaterdecies*»; al comma 9-*quinquies* inserire dopo le parole: «per ciascun consigliere», la seguente: «circoscrizionale»; - al comma 16-*quinquies*, sostituire le parole: «16-*quinquies*, primo periodo», ovunque ricorrano, con le seguenti: «del primo periodo del presente comma»; al comma 17-*quinquies*, sostituire le parole: «comma 19-*quater*» con le seguenti: «comma 17-*quater*»; - al comma l8-*quater*, sostituire le parole: «dell'evasione e» con le seguenti: «dell'elusione e»; al comma 18-*septies*, sostituire le parole: «al presente articolo» con le seguenti: «ai commi da 18-*octies* a 18-*decies*»; Alla Tabella 1, sopprimere le seguenti voci: «31 dicembre 2010 articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze 21 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta* *Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 2010».

Ogni voto di fiducia su un singolo provvedimento è in realtà una umiliazione del Parlamento e al contempo dell'opinione pubblica, che è privata del diritto di conoscere in modo puntuale ragioni e motivazioni di ogni singola norma. Non è solo questo. I voti di fiducia si succedono in modo incoerente: con il voto successivo si erode la base politica del precedente. Abbiamo avuto tra settembre e dicembre due voti di fiducia politici, a fine settembre la promessa dei famosi cinque punti per il rilancio e nulla è successo. Così come nulla è accaduto dopo la fiducia di dicembre. E da ultimo la promessa frustata all'economia, già scomparsa dalla agenda politica. Come hanno riconosciuto tutti, una frustata inconsistente, fatta di rinnovo di cambiali già firmate (il Mezzogiorno, il piano casa, la riforma degli incentivi all'economia): avreste dovuto venire qui a dire quello che avete fatto sulla base degli impegni, non certo a rinnovare le cambiali del "faremo". E poi un po' di ridicole fumisterie ideologiche: cambiare l'articolo 41 della Costituzione, quello sulla libertà economica, si può anche fare, se si riesce a scriverlo meglio; ma naturalmente non c'entra nulla con le riforme necessarie a modernizzare il Paese. Da quando è nata la Corte costituzionale, nel lontano 1956, non una sola legge liberalizzatrice è stata dichiarata incostituzionale per violazione di quell'articolo. Comunque, c'è traccia di questa volontà riformatrice nel milleproroghe? Se non una frustata, almeno una carezza di incoraggiamento alla competitività e alla crescita del Paese? Non c'è nulla, anzi le politiche presenti sono contro. I peggiori difetti della legge finanziaria rientrano dalla finestra, come l'affastellarsi di norme contraddittorie per compiacere i portatori dì piccoli interessi, una opacità dei conti. I Fondi indifferenziati introdotti nella legge di stabilità sono lo strumento della mancata trasparenza, come ha ben ricordato ieri il senatore Morando.

e il suo gonnellino da cui emergono oggetti di ogni genere, da un divano ad un servizio di piatti per 12 persone: era una sfida all'impenetrabilità dei solidi. E qui c'è l'impenetrabilità delle coperture: si finanziano nuovi interventi pescando sempre dal gonnellino dei fondi indifferenziati, ma in silenzio si definanziano altre iniziative, presentate in pompa magna come successi dell'iniziativa del Governo. I Ministri strillano che ora cambierà tutto con il nuovo articolo 41, sarà permesso tutto ciò che non è espressamente vietato. Ma nel milleproroghe, signor Sottosegretario, c'è perfino il rinvio della liberalizzazione dei bagnini. Avete paura anche dei bagnini e che si possa accedere a detta professione senza esami e controlli. Figurarsi se avrete la forza politica di aprire i mercati protetti attorno ai grandi interessi: gli ordini professionali, la filiera del farmaco, le assicurazioni, il mercato dell'energia, dei servizi pubblici e bancari, lì dove si accrescerebbe la competitività Paese e si consentirebbero vantaggi di rilievo per le tasche del consumatore.

Se capita una calamità naturale, invece di pensare a riforme strutturali, a meccanismi assicurativi e solidali, prevedete che le Regioni avranno un solo dovere: un aumento generalizzato di tasse, tributi, tariffe. Il PIL viene depresso dalla calamità e a quei cittadini ed imprese si chiede di pagare più tasse di prima. Il meccanismo di raccolta e smaltimento dei rifiuti è in crisi? Si dovrebbero immaginare vincoli per l'efficienza nella gestione, interdizione dei cattivi amministratori, lotta all'evasione della tariffa? Si rovescia il tutto e si risolve il problema con una semplice risposta: più tasse. I Comuni gestiti in modo efficiente sono impiccati al feticcio del patto di stabilità, senza alcuna autonomia di spesa anche delle risorse proprie. I Comuni che non sanno amministrare hanno mano libera nell'aumento delle tasse. Naturalmente non manca il consueto premio all'evasione. I truffatori delle quote latte hanno il loro riconoscimento con 5 milioni di euro, che naturalmente saranno molto di più con le inevitabili sanzioni europee. Ci avete parlato di un nuovo piano delle infrastrutture. Penso alla banda larga, infrastruttura informatica essenziale per la competitività delle imprese. già in enorme ritardo per la realizzazione di una prima insufficiente ossatura: stiamo lavorando su una infrastruttura come se facessimo oggi una autostrada ad una corsia,

L'11 gennaio 2011, il CIPE stanzia alcuni fondi per gli investimenti nella banda larga, con grande annuncio del Governo. Dopo pochi giorni con il milleproroghe la delibera viene definanziata ed i fondi destinati ad altra cosa. Come fanno gli investitori ad avere fiducia in un Governo che si comporta in questo modo? Con la frustata avete promesso una pubblica amministrazione più efficiente, l'alleggerimento del peso dello Stato, ma il ministro Brunetta è scomparso. Ora è vero, signor Sottosegretario, che per noi piccoli è piuttosto facile scomparire, ma con lui è scomparsa anche ogni promessa di introdurre nella pubblica amministrazione stringenti condizioni di valutazione e di riconoscimento del merito. riuscite a fare male anche le cose giuste. La previsione di 30 milioni di euro aggiuntivi per l'alluvione del Veneto è certamente una cosa giusta, una cifra che però non basta neppure a coprire tagli ben superiori fatti nel bilancio della Regione sui fondi della sicurezza idraulica. Dunque, alla fine il bilancio è che ci sono meno soldi di prima per la sicurezza dei cittadini. Si interviene per rafforzare le banche di fronte ai nuovi test per l'attuazione di Basilea 3.

ma siete sicuri che sia bene finanziare quest'operazione rendendo più costose fiscalmente le fusioni delle imprese, in un Paese in cui queste ultime andrebbero incentivate? conclusione, domenica c'è stata una grande manifestazione di indignazione collettiva non tanto per i comportamenti privati del *Premier*, ma per il loro insopportabile debordare nella sfera pubblica. Eguale indignazione vi sarà per questo immobilismo del Governo. L'Europa sta pensando ad un nuovo Patto i cui criteri fondativi saranno l'indebitamento, la produttività, la quota di fondi destinati a ricerca, infrastruttura ed educazione. Siamo indietro su tutti e tre i parametri. Ci sarebbe bisogno di un grande sforzo collettivo stimolato dalla buona politica. Il Governo preferisce non sentire, non vedere, non agire.

cosiddetto milleproroghe, che faceva acqua da tutte le parti. La fiducia è quella degli italiani verso il Governo, come quella dei consumatori e dei risparmiatori verso le banche. Questa fiducia viene posta invece per assecondare gli interessi dei grandi potentati economici, in special modo dei banchieri. La fiducia degli italiani verso il Governo si riduce, a riprova che mettere nel maxiemendamento i *desiderata* di lorsignori può risultare controproducente.

emendamenti tendenti a dare l'ennesimo aiuto ai lorsignori banchieri. Qualche giorno fa, quando il governatore della Banca d'Italia Draghi (si dice che sia candidato alla Banca centrale europea: Goldman Sachs andrà alla BCE) buona parte del direttorio della Banca d'Italia sono andati con il cappello in mano a Piazza del Gesù, sede dell'ABI, per partecipare all'esecutivo di quell'associazione, puntini puntini, avuto la certezza che dovevano essere concertate misure salvabanche, oltre alle migliori disposizioni, spesso fraudolente, per piazzare obbligazioni bancarie in scadenza. ci sono circa 230 miliardi di euro di obbligazioni bancarie che i risparmiatori non vogliono. I risparmiatori, già scottati

Ed è proprio quest'ultimo rapporto che ha fotografato un risparmiatore scettico e disincantato rispetto alla capacità delle banche di contribuire allo sviluppo dei nuclei familiari, delle aziende e, più in generale, della crescita dell'economia. Gli istituti di credito risultano infatti avidi, arroganti, menefreghisti ed inaffidabili, soggetti detestati e detestabili. In

effetti, non solo chiedere denaro in prestito alle banche, ma anche la più semplice delle operazioni bancarie - come cambiare un assegno bancario o circolare di poche centinaia di euro presso lo sportello in cui è tratto e radicato il conto corrente - diventa una missione impossibile, perché le banche devono lucrarci,

cambiare contanti allo sportello, impongono al cliente di versare l'assegno sul conto corrente, in modo da poterci lucrare le commissioni di versamento e di prelievo, i giorni di valuta, oltre ad evitare qualsiasi rischio.

ha indicato un netto peggioramento perfino della situazione economica individuale degli ultimi anni, che legato alla tracotanza e alla vessatorietà dei contratti,

poca o nessunissima fiducia nelle istituzioni creditizie; ma voi - ripeto - fornite loro un aiutino, praticamente sotto diretta dettatura dei banchieri degli emendamenti che dovrebbero davvero riferisco in particolare alle disposizioni per il sistema bancario, alla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative a svalutazioni di credito non ancora dedotto dal reddito imponibile, ai crediti d'imposta.

forse devono pagare quei 40 milioni di euro elargiti a banchieri che se ne sono andati dopo aver distrutto qualsiasi fiducia. La cosa che ci fa

2010. I risparmiatori, le associazioni, i correntisti che si ribellano ai banchieri vanno alle Sezioni unite di Cassazione, ottengono sentenze, e voi fate il colpo di spugna sui diritti. Voi, Governo, che avete già assecondato i *desiderata* dei banchieri con lo svuotamento della *class* *action*, di quello strumento che in un mercato non in un feticcio di mercato - è indispensabile per dare la certezza del diritto e dare degli strumenti di difesa al popolo dei consumatori. Questa sentenza aveva posto la definitiva pietra tombale sulle diffuse illegalità bancarie in merito all'usura legalizzata, denominata anatocismo: gli interessi capitalizzati trimestralmente.

chiude il conto corrente. E voi invece inserite in questo decreto una norma *ad hoc* per cancellare i diritti delle piccole e medie imprese taglieggiate dalle banche. taglieggiate dalle banche. Noi dell'Italia dei Valori continueremo a stare dalla parte della povera gente, voi continuate ad andare a braccetto con i banchieri. E vedrete che vi troverete molto bene, in buona compagnia. Ma state certi che, come in passato sono state portate davanti alla Corte costituzionale norme che cancellavano i diritti e la Corte costituzionale le ha cancellate, anche questa volta verrà portato davanti alla Corte costituzionale un vergognoso decreto salvabanche che cancella i diritti di milioni di consumatori «usurati», vessati e tartassati. apre una nuova finestra"). Colleghi, vi informo che assistono ai nostri lavori gli studenti dell'Istituto tecnico commerciale «Valentino De Fazio» di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, ai quali diamo il benvenuto*.

non ci sia bisogno di ricorrere a motivazioni esogene a questa Aula - mi riferisco al rinvio a giudizio del Presidente del Consiglio -per motivare il nostro voto contrario alla richiesta di fiducia, anche se proprio questa coincidenza (chiedere la fiducia, cioè portare il provvedimento all'interno di un ragionamento più generale sull'opera del Governo) richiederebbe forse una pausa di riflessione, una comunicazione del Presidente del Consiglio all'Aula, non essendo un fatto così usuale quello che è accaduto oggi, per quanto il nostro Paese sia abituato a molto. Quindi, anche se forse basterebbe dire «ma quale fiducia e a chi?», cercherò di stare nel merito del provvedimento e di svolgere pienamente, anche in questa occasione, la mia funzione di senatore. Intanto sul ricorso alla fiducia e a proposito del «Governo che governa», secondo il mantra che ci viene riproposto da esponenti della maggioranza in tutte le circostanze: siamo alla trentasettesima richiesta di fiducia dall'inizio della legislatura e, se togliamo le quattro richieste sui documenti politici, quindi le richieste di fiducia in senso proprio, politico, scendiamo a 33, che corrispondono più o meno ai mesi della nostra legislatura, che sono 32. Togliendo le pause per le vacanze, sono

Il ricorso al maxiemendamento in sostanza annulla il lavoro fatto dal Parlamento, quasi sempre per modificare non solo il testo uscito dal lavoro parlamentare, ma lo stesso testo originario Se si tratta di decreti, teoricamente adottati per necessità e urgenza, questi testi già eterogenei, di dubbia rispondenza al dettato costituzionale, vengono ulteriormente - diciamo così - arricchiti di materie estranee.

della trasparenza del dibattito in Commissione e del maxiemendamento presentato dal Governo, che non annulla il lavoro fatto dalla Commissione; ma ciò non toglie che le

L'ultima, e forse la più creativa, è quella della delegificazione tramite decreto‑legge, ovvero ciò che questo milleproroghe produce nell'articolo 1, comma 2, poi modificato (sul «Non si può immaginare di delegificare con decreto‑legge, spostando il potere di disciplina dal Parlamento al Governo e, ancor più, non si può parlare di necessità e urgenza in un modulo di proroga-*bis*, a sequenza di stadi, individuando il primo di essi

che sono rinviati alla discrezione assoluta del Governo, che potrà modificarli. Ho già detto che su questo punto c'è stata una correzione, dopo un ampio dibattito in Commissione, ma essa non può essere considerata sostanziale, perché

parlamentari e la gerarchia delle fonti, quindi il principio di legalità. E così il recupero - attraverso il milleproroghe - della abbandonata finanziaria, dopo avere approvato la legge di stabilità, è completato, perché se oltre a far diventare *omnibus* il milleproroghe di fine anno introduciamo principi di delegificazione e comunque principi che sottraggono al Parlamento, dando loro valore di legge, le norme contenute in tale decreto, a questo punto ricostruiamo,

Infatti, andando a "spulciare" nel testo (uso questo termine perché è una tale congerie di norme che il ministro Calderoli giustamente non si fa vedere, perché altrimenti, come Ministro della semplificazione, dovrebbe votare contro), troviamo alcuni aspetti assolutamente preoccupanti. Per esempio, mi riferisco all'ex emendamento del relatore

dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione e di un corpo ispettivo autonomo e indipendente. Non sappiamo come e perché, non sappiamo altri criteri: sono solo titoli. Tutta Tutta questa materia, che sarebbe quella su cui questa maggioranza e questo Governo ogni giorno dicono di impegnarsi, con un colpo di mano, signora la stiamo affidando interamente ad un regolamento del Ministro che né quest'Aula né la Camera vedranno mai più. Per l'insieme di queste ragioni, oltre che per la mancanza totale di fiducia in questo Governo, che dovrebbe viceversa andarsene, voterò contro.

cui come esponente della maggioranza sono allineato, le ritrovo pienamente anche all'interno del provvedimento in approvazione, che è stato ampiamente esaminato nelle Commissioni 1a e 5a, che che hanno apportato significative modificazioni e, quindi, incrementato la portata del decreto stesso, in considerazione che l'oggetto lo consentiva. Per ciò che concerne l'articolo 1, si evidenzia che il decreto-legge in esame adotta una tecnica legislativa inconsueta, che si discosta da quella utilizzata nei precedenti decreti milleproroghe. In effetti, tali decreti utilizzavano commi che si avvalevano sia della tecnica della novella (ossia della modifica testuale di atti legislativi previgenti) sia della proroga dell'efficacia temporale, senza peraltro modificare formalmente le disposizioni vigenti. Per contro, l'articolo 1 in esame fissa, al comma 1, un nuovo termine, il 31 marzo 2011, per 63 disposizioni previgenti inserite nella tabella 1 del provvedimento al comma 2, rimette al Governo la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici relativi a tutti i provvedimenti elencati nella tabella 1. In particolare, il comma 2 autorizza il Governo a modificare, con una fonte secondaria, il termine di vigenza di normative contenute in fonti di rango primario. Su tale aspetto il dibattito e gli emendamenti discussi in Commissione hanno consentito di coinvolgere il Parlamento nella definizione delle proroghe, attraverso i pareri delle Commissioni competenti; in particolare le Commissioni riunite hanno approvato l'emendamento 1.268 (testo 3), il quale dispone che le proroghe di termini di cui al provvedimento in esame vengano disposte, previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario.

2011, che riprende le istanze accolte da alcuni ordini del giorno, tra i quali l'ordine del giorno a firma del senatore Latronico, del sottoscritto e di altri colleghi per il ripristino dei fondi per il 5 per mille, accolto dal Governo nell'ambito della discussione relativa al disegno di legge Atto Senato n. 2464. La dotazione del fondo, che era pari a 200 milioni di euro, viene aumentato fino all'ammontare di 400 milioni di euro. Tale importo è comprensivo della quota di 100 milioni di euro destinata a interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, Lo stesso decreto nel testo originale contiene delle norme molto importanti, tra le quali ricordiamo gli interventi di salvaguardia della stabilità finanziaria dell'euro.

per pervenire alla definizione del contenzioso ancora aperto riguardante i lavori, le forniture e gli espropri connessi ad alcune opere realizzate per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali «Torino 2006» In fase di discussione ed esame in Commissione tale termine è stato prorogato, a seguito di un emendamento sottoscritto da me e dalla collega Boldi, fino al 31 Con l'esame in Commissione, inoltre, si sono date risposte concrete alle questioni riguardanti l'Abruzzo, introducendo un pacchetto di norme per i terremotati. In particolare, viene stabilito rinvio al 1° novembre della restituzione delle tasse per i Comuni colpiti dal terremoto, la proroga della cassa integrazione per i lavoratori della Finmek e l'autorizzazione al comune dell'Aquila e ai Comuni montani del cratere sismico di assumere per i prossimi tre anni personale a tempo determinato con una spesa massima di un milione di euro. Relativamente al blocco degli sfratti, viene prorogato di un ulteriore anno (dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011) il termine per le categorie disagiate. al 31 dicembre 2013 il biglietto del cinema subirà un aumento di un euro. Con le risorse incassate si potrà finanziare la produzione cinematografica nazionale (il Governo pensa di incassare 45 milioni nel 2011 e 90 milioni per i due anni successivi). Per le Regioni alluvionate, al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, vengono stanziati nuovi fondi per le calamità per una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Infine, viene stabilita la possibilità per le Regioni colpite da calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, nel caso in cui non riescano a coprire le spese della ricostruzione, di aumentare i tributi, le addizionali, le addizionali regionali e anche l'imposta regionale sulla benzina.

la proroga per un ulteriore biennio (2011-2012) per l'utilizzo dei disavanzi di amministrazione risultanti dai propri bilanci 2007 e 2008 relativi alla gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como allo scopo di fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi pubblici di navigazione lacuale relative agli esercizi 2011 e 2012 garantendone così la continuità. emendamento ha trovato la concordia dei Gruppi di maggioranza, costituisce una risposta importante per le esigenze del turismo dei laghi e avrà ricadute positive per l'occupazione. Altri emendamenti di mia iniziativa hanno trovato accoglimento, essendo stati assorbiti da emendamenti presentati molto opportunamente dai relatori, anche a seguito dell'ampio dibattito svolto dalle Commissioni riunite 1a e 5a, e inseriti nel maxiemendamento alla nostra attenzione. In particolare, voglio segnalare la modifica al comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 che rivede per gli anni 2011 e 2012 il limite fissato per la contrazione dei mutui da parte dei Comuni fissandolo rispettivamente al 12 per cento e al 10 per cento e, quindi, accogliendo una istanza particolarmente auspicata dai Comuni, soprattutto per quelli sotto i 5.000 abitanti. È stato altresì affrontato il tema inerente all'obbligo della dismissione delle partecipazioni azionarie dei Comuni con meno di 30.000 abitanti. Tale argomento aveva già trovato attenzione nell'ambito della legge di stabilità non risolvendo del tutto le criticità poste dai Comuni. L'emendamento approvato porta opportunamente il termine al 31 dicembre 2013, e fa salve dalla dismissione le società che conseguiranno un bilancio attivo nel triennio. Da ultimo, mi vorrei soffermare sull'esigenza da parte del Governo di affrontare, così come è stato risolto il tema delle quote latte, l'argomento inerente al finanziamento da destinare all'Associazione italiana allevatori, associazione che opera nel settore della genetica e che impiega 2.500 persone addette al controllo, alla promozione del miglioramento genetico della zootecnia e alla sicurezza alimentare. In effetti, il finanziamento nell'esercizio 2010 era pari a 62 milioni di euro, l'ipotesi di riduzione era di 25 milioni di euro ed essendo attualmente senza previsione di copertura finanziaria, auspico che in un prossimo provvedimento possa essere ripristinato. Per le ragioni appena esposte, che hanno consentito un netto miglioramento del decreto presentato alla nostra attenzione, che include, appunto, gli emendamenti approvati nelle Commissioni competenti, ritengo che il Governo debba continuare a godere della fiducia del Parlamento.

è una fiducia ampiamente annunciata, perché da subito il decreto milleproroghe è diventato un campo di battaglia in cui la maggioranza si è scontrata o accordata, di volta in volta, sulle questioni elettoralmente sensibili, e non altro. L'agricoltura è diventata la rappresentazione più evidente di tutto questo: lo specchio fedele di come questo Governo sta operando. Improvvisazione, ricatti reciproci, zero programmazione, zero senso di responsabilità: in agricoltura è esattamente questo lo scenario. Una serie di comparti che attendono risposte e che sono in emergenza. I dati li ha forniti ieri, in modo puntuale, la collega Bertuzzi, e non li ripeterò. Il settore ittico, la filiera del bieticolo per la produzione di zucchero, la zootecnia e il controllo della qualità, le produzioni in serra e l'insostenibile costo del gasolio, il problema dell'esposizione debitoria nei confronti dell'INPS, che sta mettendo in ginocchio le aziende agricole, in particolare del Sud, non sono parole d'ordine o titoli vuoti, ma problemi reali di centinaia di aziende reali. Sono migliaia di persone che vivono di questo, che sono appese a promesse mai mantenute e non sanno se proseguire l'attività o arrendersi e chiudere le proprie aziende. Ogni volta si rinvia al successivo provvedimento e la volta successiva la risposta è sempre una sola, e sempre la stessa: non ci sono risorse. Non ci sono risorse per accompagnare le riconversioni imposte da nuove esigenze di competitività internazionale e da adeguamenti dovuti ai parametri europei; sono risorse per attenuare costi di produzione in continuo aumento, che causano un continuo calo di redditività per le aziende. Le risorse ci sono solo per un'unica missione: il non pagamento delle multe delle quote latte. È una vergogna! Avevate provato il colpo grosso dei 30 milioni, ma era troppo anche per voi; l'avete ridotto a 5 milioni, *in extremis*. Sì, le risorse sono diminuite, ma la sostanza non cambia e neppure l'obiettivo. Di proroga in proroga, state predisponendo la sanatoria finale per gli splafonatori. Del resto, è la missione che la Lega ha dal primo giorno in cui si è insediata, la ragione per cui non voleva abbandonare il Ministero delle politiche agricole, la ragione per cui presidia costantemente il Dipartimento dell'agricoltura e detta legge al Ministro in carica. Vorrei poter trasmettere a quest'Aula la rabbia e la mortificazione delle tante aziende che si sono indebitate per mettersi in regola; migliaia di aziende, cariche di rate pesanti che hanno sostenuto per onorare il debito, che continuano a subire la concorrenza sleale di chi continua a produrre fuori da ogni regola. È difficile ricordare un Governo così spregiudicato con il settore agricolo, come questo. Nessuna programmazione, un *escamotage* dietro l'altro, con situazioni che arrivano al grottesco: un Ministro delle politiche agricole che accenna proteste in solitudine, nel disinteresse generale del suo Governo e della sua maggioranza. Mentre il Ministro dichiara tutto il suo sdegno e la sua contrarietà al rinvio dei pagamenti delle quote latte e ne dichiara l'illegittimità, mentre dà rassicurazioni a mezzo stampa che le regole trionferanno, il suo Governo e la sua maggioranza vanno esattamente in senso contrario: dicono sì alla proroga di ulteriori sei mesi e dimostrano, con scelte concrete, che la questione quote latte è tutt'altro che chiusa, in spregio alle sanzioni preannunciate da Bruxelles. Allora, mentre invitiamo il Ministro delle politiche agricole a riflettere seriamente sul senso del proprio ruolo e della propria autorevolezza, non smetteremo mai di dire a questo Governo, ancorché in agonia, e vogliamo dirlo al ministro Tremonti direttamente, che se una ripresa può esserci, se una crescita può ripartire in questo Paese, l'agricoltura può determinare una parte importante di questa crescita, perché ha vocazioni vere, ha materia prima, dispone, più che altri settori, di *know-how* inediti e preziosi, ma ha bisogno di politiche non di *boutade*; ha bisogno di dotazioni finanziarie che mettano in condizioni le aziende di ripartire, di costruire sistemi efficienti organizzati, per andare sui mercati internazionali. Investire sull'agricoltura oggi è scelta lungimirante, è di prospettiva, è di futuro; ci sono spazi, mercati e clienti che emergono. L'hanno fatto la Germania e la Francia; ci hanno creduto in questi due anni di crisi acuta del sistema agricolo. però la convinzione che l'agroalimentare è questione centrale e non residuale. Serve autorevolezza del Governo in Europa per stringere alleanze forti con altri Paesi, perché nelle politiche comunitarie siano determinanti e premiati fattori come la qualità, l'efficienza, la sostenibilità ambientale ed economica, la tecnologia e l'organizzazione, l'etica nel lavoro, a cui deve tendere questo nostro Paese per far emergere davvero il *made in Italy*. Ma è un appello che sappiamo che cade nel vuoto, perché state andando esattamente nel senso opposto. State brillando per assenza e insipienza; state tagliando addirittura i rami più forti su cui siamo appoggiati: i sistemi di controllo della qualità, accompagnando il tutto con un'insopportabile demagogia e populismo. Festeggiate e brindate all'etichettatura tutta italiana e intanto state radendo al suolo il sistema di controllo della zootecnia italiana. Avete azzerato, senza batter ciglio, il fondo per il funzionamento delle APA, i centri territoriali di controllo per il patrimonio zootecnico, per il miglioramento genetico. Dal 1° gennaio 2011 nessun sostegno pubblico ci sarà. Dunque, migliaia di aziende agricole senza assistenza, oltre 2.000 addetti, professionisti capaci, competenze preziose, che a giorni saranno senza occupazione. Abbiamo cercato una soluzione fino all'ultimo minuto, non una difesa ad oltranza del sistema esistente. Abbiamo proposto una riorganizzazione delle APA, ottimizzazione dei costi, aggregazione di servizi. Abbiamo proposto di destinare almeno 25 milioni di quel fondo per permettere un'organizzazione nuova, di trovare una soluzione assieme alle Regioni, assieme agli stessi produttori. Avete rigettato anche questo, e non avete avanzato nessuna altra ipotesi. Concludo dicendo anche che questa non deve apparire solo come questione di settore. Stiamo parlando di sicurezza alimentare, di metodi di controllo rigorosi, che costituiscono i fondamenti della garanzia sulla qualità degli alimenti per i consumatori e la loro salute. Deve essere chiaro che con tali omissioni stiamo smantellando un sistema; lo dico alla maggioranza che si appresta ad approvare questo, se non fosse sufficientemente chiaro, e dovrà renderne conto. devono sapere che la questione quote latte non è solo una vicenda agricola, è anche affar loro. I milioni di euro di multe non pagate dai grandi produttori li stanno pagando tutti i cittadini, ognuno in quota parte; e la copertura di questa operazione, ancorché ridotta con un taglio lineare dei fondi di tutti i Ministeri, si traduce concretamente in tagli ulteriori ai fondi per il sociale, per il diritto allo studio, per il presidio dei territori, per la sicurezza, per i Corpi di polizia. Dunque, è affar loro e dell'intera società. Altro che fiducia! Fate presto a staccare la spina, prima che le macerie che state lasciando siano insormontabili.

alcune delle più desolanti riguardano aspetti legati alle politiche ambientali. Parlerò brevemente soltanto di una di esse, ossia la

dalla Camera dei deputati, che osservò due aspetti metodologici di assoluta evidenza: il primo è che una legge non può intervenire su una sentenza passata in giudicato, come è il caso delle ordinanze di demolizione degli immobili abusivi disposte dalla magistratura in Campania; il secondo aspetto è che non si possono fare leggi *ad regionem*. Anche se siete abituati a fare leggi soltanto per singoli cittadini, non eravamo ancora abituati alla pratica delle leggi riservate soltanto a una parte del territorio nazionale. In questo milleproroghe, quindi, da una parte si tagliano i fondi straordinari stanziati a suo tempo da questo Governo per la lotta al dissesto idrogeologico (da 900 milioni a 800 milioni), e dall'altra si dà una bella mano ad incentivare, ad incoraggiare l'abusivismo edilizio. Come si sa, la Regione Campania tra le Regioni italiane, quella che ha pagato il prezzo più pesante, più alto all'abusivismo edilizio. Come si sa, l'abusivismo edilizio, in Campania come altrove, vede spesso il coinvolgimento diretto **(ore 18,30)** (*Segue* DELLA SETA). Come si sa, l'abusivismo edilizio è una delle principali cause che rendono il territorio italiano insicuro, e che poi ogni anno trasformano eventi metereologici più o meno eccezionali in tragedie con morti e feriti.

legge, e dà una bella spinta a rendere il territorio, in questo caso quello della Campania, sempre più fragile e insicuro per chi ci vive. L'intendimento, esplicito anche nelle nelle dichiarazioni di chi ha proposto un emendamento approvato dalle Commissioni riunite e recepito dal Governo nel maxiemendamento, è che questa norma sia una sorta di premessa alla riapertura dei termini del condono edilizio del 2003 per la sola Campania. Ci troviamo nuovamente di fronte ad una norma *ad regionem*. Insomma, quella che voi avete inserito in questo caso è davvero una norma che penalizza la legalità, la qualità la qualità del territorio e soprattutto rende più insicura la vita di tutti quegli italiani che abitano in case sorte dove non si sarebbe dovuto costruire, in zone

e di Ischia. Voi il regalo che fate alla Campania è quello di dare una bella spinta in questa stessa direzione. Complimenti. *(PD)*. Signora Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, inizialmente mi soffermerò sulle problematiche inerenti al tema dell'agricoltura, rifacendomi all'intervento di grande spessore, che tanti di noi profondamente condividono, della collega Pignedoli e interpretando l'avviso dei colleghi del Gruppo del Partito Democratico in 9a Commissione per manifestare ancora una volta, l'ennesima, il nostro forte dissenso sul provvedimento in esame, anche ad esito dei contenuti di questo maxiemendamento di cui in questo pomeriggio discutiamo. La delusione è tanto più rilevante quanto più si pensi alle innumerevoli circostanze in cui il Governo, in Commissione e nell'Aula del Senato, così come il Ministro precedente e il suo successore in varie occasioni pubbliche passate e recenti attraverso dichiarazioni in convegni, interviste ai mezzi di informazione radiotelevisivi e della carta stampata, ha assunto impegni precisi rinviando al successivo provvedimento utile la risposta alle varie ed urgenti questioni sul tappeto. Quello del decreto milleproroghe è un altro appuntamento clamorosamente mancato. Questa volta però c'è di più, non soltanto perché a circa tre anni dall'inizio della legislatura si conferma la più totale disattenzione e, anzi, l'assoluta sordità del Governo, in particolare del Ministro dell'economia, verso le antiche e recenti sofferenze del settore primario, ma anche perché nell'ultimo periodo abbiamo dovuto anche ascoltare proclami da parte del ministro Galan che ci ha dipinto uno scenario per l'immediato futuro apparentemente assai incoraggiante. Sta di fatto, però, che quella prospettiva non si è realizzata con i provvedimenti finanziari di fine 2010 (Decisione di finanza pubblica e legge di stabilità), né prende corpo e forma oggi attraverso il decreto di proroga termini che, pur tuttavia, trova il modo di occuparsi nuovamente degli splafonatori delle quote latte. Ho seguito la gran parte dei lavori delle Commissioni riunite 1a e 5a la scorsa settimana; conoscevo la prima formulazione dell'emendamento sulle quote latte e ho preso visione della seconda, per la quale la copertura finanziaria è stata mutata cedendo al solito espediente del taglio lineare. Oggi troviamo un terzo cambiamento nella copertura, ma quel che più si nota è il drastico taglio

perché allora quello sproposito di 30 milioni? Mi chiedo a cosa sarebbero serviti, signora Presidente. Potrei ricorrere ad una celebre frase molto abusata: «A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si indovina». Non dico altro; semmai penso, ma non dico.

ad altri piani di azione agricoli come, per esempio, il fondo per lo sviluppo agricolo, il che rappresenterebbe un danno incalcolabile per tutta la filiera agroalimentare e per il settore agroindustriale collegato. Farlo attraverso un emendamento del Governo sul quale è posta la questione di fiducia è ancora più stridente; suona quasi come un atto di sfida alle istituzioni europee. Devo dare atto al ministro Galan di aver fatto squillare il campanello d'allarme. Ho visto circolare nei giorni scorsi una lettera durissima

parere assolutamente contrario" (sottolineati ed in neretto) all'emendamento, citando tra l'altro la formale diffida del commissario Ciolos, della quale avevamo avuto da tempo notizia, dal luglio passato,

e il Ministro non si dimise. Mi pare allora che "la storia si ripeta" anche nella circostanza del milleproroghe; magari in modo meno eclatante e clamoroso, ma si ripete. Non parliamo poi del fondo bieticolo-saccarifero, per il quale non è previsto alcunché, malgrado le assicurazioni rese dal Ministro durante l'audizione del 28 luglio svolta in Commissione agricoltura. il ministro Galan preannunciò - leggo testualmente dal resoconto stenografico di quella seduta - «un pacchetto di misure per rispondere alle esigenze indifferibili dell'agricoltura italiana», all'interno del quale sarebbero rientrati - aggiungo e leggo ancora testualmente - «interventi a favore del settore

Quanto al resto, il Ministro dichiarò testualmente: «Gli altri 65 milioni sono contemplati nel pacchetto di provvedimenti previsto e sarà il primo impegno che dovrà essere assunto». essere assunto». Ma mi pare che quell'impegno non sia stato ancora neanche accennato, e non dico mantenuto o garantito. Per AGEA, in compenso, c'è la proroga degli incarichi dirigenziali, una bella soddisfazione. Sono rimaste invece inascoltate tante altre nostre proposte, sempre restando in tema di proroghe e dunque in coerenza con la natura e lo spirito dello strumento di cui oggi oggi discutiamo, il milleproroghe. Mi riferisco, ad esempio, al credito di imposta per l'internazionalizzazione in agricoltura; alle agevolazioni per il gasolio occorrente al riscaldamento delle coltivazioni sotto serra; al sostegno all'impresa giovanile e femminile in agricoltura; all'ICI sui fabbricati rurali, cioè su quegli immobili che, pur essendo utilizzati

Niente ancora su tutto questo. I nostri emendamenti puntualmente sono stati respinti. Aspettiamo magari il solito annuncio che ci dirà: «Alla prossima occasione utile...», eccetera, eccetera, come è avvenuto in passato.

Per concludere, sul tema agricoltura, un tema così delicato, non abbiamo rilevato alcunché, niente da parte del Governo, a parte qualche piccola cosa che abbiamo testé che abbiamo testé individuato. A queste necessità, alle varie esigenze rappresentate, il Governo non risponde. Il Governo va in soccorso a qualche decina di splafonatori in un'area geografica del Paese ben definita e limitata, e non si trovano invece 25 milioni per garantire a 20.000 ‑ dico 20.000 ‑ aziende zootecniche, che soffrono una situazione di grave difficoltà, di mantenere lo *standard* di controlli seri ed attendibili sul patrimonio zootecnico. Mi pare che la misura sia colma e questo sia praticamente rilevabile...

un diniego da parte del Governo sulla programmazione negoziata, sui patti territoriali, sui contratti d'area e sugli strumenti di sviluppo. Dunque, si ha la sensazione di una letterale falcidia, effetto - presumo - di un disegno preordinato che non è sintomo di rigore, ma di rigidità che è, per l'appunto, il contrario

parzialmente. Ne prendiamo atto, signora Presidente, così come prendiamo atto di una copertura finanziaria sbagliata che toglie soldi alla Campania e li ridà con la stessa mano alle zone colpite colpite dall'alluvione del novembre scorso. Anche questo atteggiamento del Governo è molto grave ed offre il senso e la misura della superficialità con cui questo provvedimento e questo strumento sono stati attivati.

la seduta pomeridiana di oggi sarà tolta a conclusione della discussione generale. Le dichiarazioni di voto avranno luogo nella seduta antimeridiana di domani, anticipata alle ore 9. Seguirà quindi la chiama sulla fiducia, che Seguirà quindi la chiama sulla fiducia, che avrà inizio intorno alle ore 10. Avverto inoltre che, come già comunicato per le vie brevi ai Gruppi, l'informativa del Governo sugli sbarchi di clandestini a Lampedusa si svolgerà in altra data, al fine dell'acquisizione di maggiori elementi informativi. alcuni dati saranno forniti già domani nel corso dell'informativa del Ministro degli affari esteri - fissata per le ore 16 - sui più recenti sviluppi della situazione nei Paesi del Mediterraneo.

voglio ricordare qui che qualche anno fa il presidente Ciampi ritenne, in ragione della diversità profonda tra il testo originariamente presentato e quello alla fine pervenuto,

avere sott'occhio la testimonianza diretta e difficilmente discutibile del fatto che la congiunzione tra la prassi del decreto-legge, del maxiemendamento e della fiducia di fatto costituisce un avvilimento sistematico ed ontologico del lavoro parlamentare. Il decreto-legge sin dall'inizio contrae e schiaccia la possibilità di discussione. Si sottosta ad una sorta di

Ciò determina una forma di autocensura del parlamentare e dei Gruppi parlamentari ed invita ad una sorta di concertazione sotto ricatto. potrebbe anche essere un ricatto positivo, a buon fine, per riuscire a produrre un testo che abbia una finalità riconoscibile ed un'efficacia nei fini,

(cosa che di per sé era già discutibile, trattandosi di una condizione limitativa, nel senso che bisognava accettare una sorta di autoconsapevole limitazione), ma arriva in fondo interpolato dal maxiemendamento finale. Non solo: questo maxiemendamento finale è contrassegnato da una specificità funzionale. Infatti, se è vero che all'inizio, nel giudizio di ammissibilità, una severa scrematura degli emendamenti aveva escluso tutti quelli che non avevano una finalità di proroga, di proroga, oggi ritroviamo nel testo finale del maxiemendamento una quantità di disposizioni che ben poco hanno a che vedere con la proroga. questo si ricava che Senato e Camera, le Assemblee elettive e responsabili dell'attività legislativa,

bisogna aggiungere che questo stesso destino è replicato in modo perfetto anche per l'Aula della Camera, che riceverà questo testo e dovrà affrettarsi ad approvarlo senza discutere, perché non ne avrà materialmente il tempo, come del resto noi non abbiamo avuto il tempo oggi di considerare le modifiche introdotte dal maxiemendamento perché ci sono stati concessi soltanto pochissimi minuti. tutto questo in nome di che cosa? Per contraddire l'adagio, la vulgata che l'attuale Governo ripete continuamente, vale a dire: «Non metteremo le mani nelle tasche degli italiani», in realtà, all'interno di questo maxiemendamento ci sono imposte aggiuntive; c'è un aumento di spesa per motivi vari che non ha giustificazione; c'è, al contrario, un mancato sostegno a settori essenziali della società, che invece vengono depauperati e privati di risorse; c'è, alla fine, la moltiplicazione dell'illegalismo.

aumento dei costi della politica. Dopo tutti i discorsi retorici che abbiamo ascoltato in quest'Aula, viene lasciata la possibilità di aumentare il numero degli assessori e dei consiglieri nelle grandi città; viene accresciuto l'incremento di indennità; c'è poi - cosa forse ancora più grave - un ribaltamento del rapporto tra legislazione giurisdizione. Il fenomeno degli abusi edilizi in Campania è il più rilevante tra tutti, ma in questo caso assistiamo ad una sospensione di effetti di sentenze penali di condanna, anche definitive, che

l'espressione - che è addirittura involontariamente ironica, perché si sostiene che il ripensamento sulla demolizione degli abusi edilizi si rende necessario per permettere alle autorità preposte di condurre una matura riflessione sui nuovi assetti paesistici. La Consulta, che aveva trattato questo argomento, sarà

prendere supplenti soltanto all'interno della Regione ed impedire che i supplenti venissero anche da altre Regioni, era stata rigettata dalla Consulta con la massima semplicità. Senza pudore,

Particolarmente indicativo della temperie culturale in cui ci troviamo è il fatto che viene modificato il rapporto tra televisione e giornali. In Italia si vive come tutti sanno una condizione che è sconosciuta in qualsiasi Paese civile: il proprietario massimo delle reti private è è titolare del potere politico e in quanto tale è il controllore massimo delle reti pubbliche. Ma questo non gli basta! E' riuscito ad aggirare anche la norma che stabiliva che chi ha le televisioni non può avere la stampa: non ha la stampa, ma ce l'ha suo fratello, la sua famiglia. Quindi, il veto era già aggirato nella maniera più volgare e pacchiana. Oggi, poiché la voracità proprietaria del Presidente del Consiglio non è placata da questo,

inenarrabile questione del conflitto d'interesse, ignoto in qualsiasi altro Paese democratico, sulla necessità della concorrenza, della piena trasparenza degli assetti societari e così Siamo di fronte ad un provvedimento che contiene in sé tutti gli elementi, astratti e concreti, della negazione di di un reale provvedimento significativo per la ripresa economica e la trattazione corresponsabile degli elementi della vita sociale. Tutto questo per cosa? Per dare la fiducia

da una condizione a dire poco stravagante: si trova ad essere processato il 6 aprile per reati infamanti come concussione e prostituzione minorile. Il giudizio non è ancora stato dato, ma per questo solo qualsiasi Capo di Governo del mondo civile sentirebbe la necessità di liberare la scena dalla propria ingombrante presenza, come hanno fatto già fatto Kohl, Olmert ed una quantità di altri responsabili della direzione politica dei loro Paesi. Siamo arrivati all'indicibile.

Presidente, nell'esprimere la mia contrarietà al voto di fiducia, il trentasettesimo, vorrei dire al Governo che se anche in quest'Aula raccoglierà la fiducia, il fatto politico vero è che la sta perdendo nel Paese. E lo hanno dimostrato le manifestazioni delle donne di domenica scorsa: in centinaia di migliaia le donne sono scese in piazza in molte importanti città del Paese per chiedere che ci sia un maggior rispetto della loro dignità. Colpiscono le accuse di faziosità lanciate dal Presidente del Consiglio, che evidentemente non concepisce e non accetta la libertà di espressione e la capacità delle donne di essere autonome e pensanti.

per rimuovere alcuni dei gravi limiti delle politiche dello sviluppo, che la negazione della crisi fatta per quasi due anni dal Governo ha in fondo favorito. E invece appare come un'altra occasione perduta, in particolare per un sistema salute sotto stress, per le difficoltà di rientrare dal debito da parte di alcune Regioni, per i costi e i fabbisognistandard che si vogliono calcolare senza i livelli essenziali di assistenza, per le notizie che arrivano agli onori della cronaca riguardo i tempi di attesa - che si allungano - per ottenere prestazioni specialistiche e diagnostiche e che costringono chi può, e anche chi non può, ma con un grave sacrificio, a mettere mano al portafoglio. Aumentano pericolosamente i tempi di attesa per chi si reca all'emergenza-urgenza e al pronto soccorso dei nostri nosocomi. Di recente, le associazioni dei medici e le organizzazioni sindacali di categoria hanno lanciato l'allarme per le lunghe attese a cui sono sottoposti anziani e bambini che accedono a questi servizi di soccorso, che - se ben funzionanti - possono salvare vite umane e ridurre la possibilità di danni permanenti. I pazienti, invece, stanno seduti per 7-8 ore su una sedia per la mancanza di letti, in attesa di essere E questo, badate bene, non accade solo nelle Regioni del Sud, ma anche nelle Regioni del Nord, dove si dice che la sanità è di eccellenza. Questi sarebbero i problemi da affrontare. Colpisce che invece nel testo del milleproroghe siano tutt'altre le questioni che vengono messe in evidenza,

si preveda che i dati raccolti dai centri per la procreazione assistita, invece di essere inviati all'Istituto superiore di sanità, debbano essere trasmessi al Ministero della salute. Non ci rassicura affatto la risposta

che accedono a queste prestazioni? Se l'unico scopo è controllare l'efficacia e il rispetto delle procedure da parte delle strutture che fanno la procreazione assistita,

migliore interesse del paziente e del rapporto tra medico e paziente, ma anche del Servizio sanitario nazionale, da cui questi professionisti dipendono. Ebbene, con questo decreto milleproroghe, il termine è rinviato al 2013:

milioni? Se la SLA è una malattia così grave, è possibile pensare ad un'assistenza *una tantum*? Forse perché si avvicinano le elezioni? È possibile capire come verrà distribuito questo fondo?

nel corso del dibattito svolto qui in Aula è emerso con chiarezza che questo provvedimento costituisce un ulteriore passo che il Governo deve compiere. Un passo necessario, non solo perché annualmente si ripropone l'esigenza di permettere ad alcune disposizioni normative di continuare ad esplicare la propria efficace, ma soprattutto perché le Commissioni referenti, la 1a e 5a, con un lavoro proficuo e preciso, peraltro condiviso, ancorché difficile, faticoso e macchinoso, hanno fornito alcune indicazioni all'Esecutivo che assumono una portata significativa, sia nell'immediato che nel futuro. indicazioni che sono oggetto del maxiemendamento presentato e su cui ci accingiamo a votare la fiducia. Certo, come solitamente avviene, le opposizioni cercano di evidenziare quello che non è stato fatto, quello per cui il Governo e la sua maggioranza, quella che lo sostiene fortemente, avrebbero potuto fare di più e meglio, evidenziando anche le discrasie, per così dire, formali di un provvedimento che avrebbe esondato i propri argini. Al di là del fatto che a tale proposito dovremo metterci d'accordo una volta per tutte se l'intervento delle Camere sia da auspicare o da evitare. Ieri infatti alcuni colleghi cercavano di argomentare la disattenzione che il Governo avrebbe mostrato oggi per le scelte fatte con precedenti provvedimenti. Così, ed è sintomo del peggioramento della trasparenza della gestione della finanza pubblica e della progressiva dequalificazione del bilancio pubblico, il decreto milleproroghe sottrae, secondo il senatore Morando, risorse un po' a tutti (imprese, famiglie, università non statali e Comuni) per finanziare interventi vaghi e inconsistenti. Ebbene, senza ripetere quanto già ricordato dai relatori, dai colleghi che mi hanno preceduto e dal rappresentante del Governo, che voglio ringraziare per il paziente lavoro e per l'infaticabile sostegno all'operato della Commissione, non credo possano essere ascritte a una mancanza di prospettiva le scelte effettuate con questo provvedimento, siano quelle di carattere emergenziale o no. Penso, ad esempio, alla proroga dei*voucher* per i cassaintegrati e ai soggetti in mobilità. Così come non può essere qualificata come generica o addirittura qualunquista la sensibilità dimostrata nei confronti di chi è chiamato ad affrontare gravi emergenze, siano quelle di natura fisica, senatrice Bassoli, come per esempio i portatori di SLA, una malattia tremenda sulla quale il Governo ha puntato la propria attenzione con un cospicuo e importante finanziamento, sia quelle di natura ambientale, penso agli abitanti dell'Abruzzo, della Liguria, del Veneto e della Campania colpiti dalle esondazioni e dalle alluvioni. Ma poi siamo così sicuri che questo provvedimento manchi di scelte anche virtuose? Certamente non possono non considerarsi positivi gli interventi relativi al Patto di stabilità, quello dei Comuni, e alla *governance* economica europea, che sempre di più costituisce il passaggio obbligato nelle decisioni di finanza pubblica. Così come, secondo me, grande rilevanza assumono le misure connesse ai vincoli di Basilea 3, poste al sistema bancario. Con le modalità di patrimonializzazione attuate si è inteso, in fondo, mettere in sicurezza le banche, per consentire loro di mantenere un forte rapporto con il territorio, in generale salvaguardare il risparmio e garantire alle piccole e medie imprese quei fondi che sono l'ossatura vitale della nostra economia. A proposito di risparmio, mi è sembrato che il Governo abbia dimostrato grande sensibilità nel riconoscere le perplessità espresse anzitutto dal senatore Morando, e anche da me in sede di Commissione, sull'originaria formulazione della norma relativa a Poste italiane, al risparmio degli italiani collocato nelle Poste. Nel maxiemendamento, infatti, è chiaro come questa realtà sia al servizio di un progetto importante come la Banca del Sud e a questo sia stato strettamente connesso. Vorrei anche ricordare la proroga alle fondazioni, cui storicamente partecipano banche popolari (le banche per eccellenza del territorio), che abbiamo in modo condiviso tutti sostenuto ed approvato. Quella proroga, unita all'auspicio - aggiungo io - a concludere quella modernizzazione del sistema delle banche popolari che oggi diventa sempre più urgente anche alla luce dei nuovi vincoli di Basilea 3, non deve trovarci impreparati. di una serie di elementi di priorità considerati come tali nell'agenda della congiuntura del Paese, come ricordava il sottosegretario Giorgetti stamane in Aula, tratteggiando le modifiche introdotte all'originario testo e spiegandone i contenuti e le motivazioni non solo tecniche. Tuttavia, credo che il dibattito fin qui svolto debba essere contestualizzato. Il provvedimento all'esame può essere ovviamente criticato nel contenuto e nelle forme, sebbene sia caduta la pregiudiziale formale (come ricordava ieri il senatore Baldassarri), ma per tener conto di un ambito più ampio di quello strettamente tecnico che incombe sui giudizi. Infatti, il provvedimento interviene in un momento decisamente particolare e la valutazione che le opposizioni hanno tentato di darne non può non risentire di un clima che sta sovrastando l'intero sistema politico istituzionale. In altre parole, leggendo tra le righe (ma neanche tanto), ascoltando la senatrice Bassoli prima e prima ancora la senatrice Adamo, dagli interventi svolti dai colleghi dell'opposizione mi sembra che si possano tirare le seguenti conclusioni: il provvedimento va respinto perché è il frutto di un Governo incapace di fornire al Paese risposte adeguate ai tempi, perché delegittimato da un Premier privo di credibilità. del senatore Morando di ieri in poi abbiamo ascoltato solo richieste di dimissioni. E il punto è proprio questo. Le dimissioni del Premier e, quindi, del Governo vengono chieste ormai come una specie di litania dal PD, da Vendola, da terzi poli. Un mantra, senatrice Bassoli, destinato a creare un clima politico a sostegno dell'azione "impolitica" delle procure e con un unico obiettivo: abbattere Berlusconi! Ma questo è l'obiettivo delle procure; non è detto che sia così utile alla politica, che sia anche il vostro obiettivo. Difatti non c'è alcuna chiarezza e, del resto, non vi preoccupa averla: tanto dopo si vedrà; l'importante è che non ci sia più Silvio Berlusconi. Berlusconi. Le elezioni sono più evocate che volute, senatrice Bassoli; mi sembra infatti che i detrattori lavorino alla rimozione del legittimo Governo, che invece continua ad essere sostenuto da una maggioranza stabile, allo scopo di instaurare un Esecutivo di salute pubblica, o meglio, di morale pubblica. Ma non vedo grandi morali in giro, non vedo grandi programmi e, soprattutto, non vedo programmi credibili. L'utopia di "più risorse per tutti" che continua a segnare in controluce la cifra delle vostre proposte, non trova più cittadinanza in Europa. Gli italiani che, invece, in Europa e nell'euro vogliono rimanerci, ne sono consapevoli. Il Governo Berlusconi è l'unico che possa rafforzare questa certezza! Senatrice Bassoli, mi consenta di concludere così: sia serena, questo lo sanno anche le donne italiane.

l'espressione di questo voto di fiducia, nonostante ciò che pensa la collega Bonfrisco, cade certamente in un momento di massima inopportunità politica, un momento nel quale a maggioranze costruite in Parlamento per addizioni improbabili corrisponde nel Paese un crescente dissenso per l'operato del Governo, più opportuno sarebbe dire per l'assenza di un operare significativo, utile, del Governo e cresce anche l'intolleranza crescente per l'indegnità dei comportamenti di chi lo guida. Lo sforzo di attenersi al merito del provvedimento è reso enorme dalla situazione paradossale in cui ci troviamo immersi, nel tentativo di dare dignità politica e sostanza ad un lavoro parlamentare frammentario e spesso incoerente, mentre sulla scena politica si rappresenta uno spettacolo da fine impero. Ciò nonostante, al merito ci atteniamo per dovere di mandato e per dignità di ruolo, una dignità tanto sostanziale quanto svilita. Quindi, vengo comunque a parlare dei contenuti, ma anche in questo caso non è facile rintracciare un senso, una logica, soprattutto non è facile rintracciare un indirizzo. Questo provvedimento ha ormai una funzione a tutti gli effetti politica; in esso, perciò, si dovrebbero rintracciare le priorità, le emergenze indifferibili sulle quali il Governo ritiene di dover intervenire. Ma se questo è il tema, dovremmo dire che quasi nulla è urgente, poiché prima del lavoro parlamentare il decreto era assai poca cosa: lo testimoniano i 1800 emendamenti presentati alle Commissioni, per oltre due terzi dai parlamentari della maggioranza. In materia di lavoro, poi, sembra che il Governo non ravvedesse emergenza alcuna, nonostante i tassi di disoccupazione imponenti, nonostante quel drammatico 29 per cento di disoccupazione giovanile, nonostante il permanere di migliaia di persone in cassa integrazione, nonostante l'aumento drammatico della precarietà. Prima del lavoro parlamentare, infatti, i profili lavoristici del provvedimento erano, ad esser lievi, minimalisti: proroghe di profilo amministrativo per la regolazione degli ammortizzatori nei settori non coperti, la cui "leggerezza" è misurata dal loro inserimento nell'articolo relativo alle proroghe non onerose; proroghe poste in luogo di una vera riforma degli ammortizzatori che invochiamo da due anni, peraltro non da soli, ma insieme a tutte le forze sociali delle rappresentanze del lavoro e delle imprese.

In un provvedimento che, stando ai dichiarati del ministro Tremonti, doveva essere la locomotiva della ripresa e dell'innovazione, di lavoro non ci si occupa. Un unico intervento sulla marea dei lavoratori precari della pubblica amministrazione: la proroga dei contratti dei precari operanti per il Ministero dell'interno agli sportelli e agli uffici per l'immigrazione; le persone - per intenderci che hanno gestito i deliranti *click day* del decreto flussi di quest'anno: se ne sarebbe potuto forse fare a meno? E che sarà nei prossimi giorni con la gestione dell'emergenza profughi? Se al lavoro ordinario si fa fronte con interventi straordinari e precari, è legittimo chiedersi con quali risorse umane si pensi di affrontare la straordinarietà e di straordinarietà dobbiamo parlare, purtroppo e per necessità. Di più non c'è, né per affrontare i problemi di funzionalità di scuole, ospedali, uffici per l'impiego - quelli che dovrebbero essere il luogo di intervento della *task force* per l'occupazione di questi tempi! dei servizi pubblici in genere, né per intervenire su funzioni nevralgiche nella gestione della crisi. Ne cito una per tutte: quella dei precari dell'INPS. 1800 lavoratori somministrati termine orribile, che si addice ai farmaci o alle punizioni - che lavorano da diversi anni nelle sedi dell'Istituto in tutta Italia attraverso le agenzie di lavoro, occupandosi delle pratiche pensionistiche e, soprattutto, negli ultimi due anni, di quelle relative alla gestione degli ammortizzatori sociali. Oltre 500 di costoro hanno già chiuso

Mi chiedo come l'INPS pensi di affrontare la gestione di queste funzioni. Bloccherà pratiche fondamentali per la gestione dell'emergenza sociale del lavoro e delle imprese li ingaggerà nuovamente con rapporti ancor più "precari", aggirando il vincolo - come già si sente dire - ed impegnando, comunque, in maniera ancor più discrezionale ed opaca, le risorse pubbliche? Pensando alle persone non si può poi ignorare che si tratta, per la stragrande maggioranza di giovani e di donne, quelle donne e quei giovani che da mesi animano la protesta nel Paese, che domenica hanno pacificamente invaso l'Italia, che chiedono lavoro, dignità, civiltà. Con loro migliaia di altri, colpiti dai tagli tremontiani, persone che, avremmo detto un tempo, dovrebbero sentire l'orgoglio di servire lo Stato, di operare per il buon funzionamento della macchina pubblica, a servizio del pubblico Come si può immaginare che questa responsabilità venga assunta, se ad essa non corrisponde un minimo riconoscimento di dignità, la possibilità di sentirsi parte di quello Stato che si deve servire? Nessun ripensamento nemmeno sugli interventi draconiani della manovra di luglio in materia di previdenza, alcuni dei quali interverranno, al di là del merito e delle loro conseguenze sociali, anche

sostenendone il diritto alla tutela e, al tempo stesso, la decisione consapevole. Non possiamo non rilevare, però, come questo importante risultato, utile anche a normalizzare un contenzioso parossistico che la scadenza così ravvicinata aveva incentivato, sia stato conseguito contro la volontà del ministro Sacconi, che ancora una volta ha ha anteposto l'attaccamento ideologico alle proprie posizioni alla tutela dei diritti dei lavoratori e, perfino, al buon senso. Per questo piena sfiducia, ministro Sacconi, a lei e al suo Governo. Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il provvedimento di proroga di termini, meglio noto come provvedimento milleproroghe, domani in approvazione, costituirà probabilmente, in una rilettura *a posteriori*, una pietra miliare dell'agonia di questa legislatura. un provvedimento che è la rappresentazione perfino grottesca di una legislatura che si era aperta all'insegna di una volontà costituente, per propositi elettorali e forza dei numeri parlamentari, ma che si è poi ritrovata a fare avanspettacolo in una situazione paradossale, in cui il verosimile è più credibile del vero e dove la stessa realtà supera ogni tipo di immaginazione. Si potrebbero sprecare infinite metafore e allegorie prendendo a pretesto i fatti, veri o presunti, che dominano la scena da mesi sui media e che ammorbano l'opinione pubblica, arrivando a condizionare inevitabilmente anche la nostra inattività. Per economia di tempo, prenderò ad esempio emblematico di questa fase politica una singolare vicenda che si è consumata in luoghi altri da quelli dovuti e che ci ha visto un po' tutti più o meno ignari spettatori, al massimo comparse, ma non attori protagonisti, come invece prerogative costituzionali avrebbero imposto. Si tratta di una questione che riguarda uno fra i settori più strategici del nostro Paese, incredibilmente e inspiegabilmente finito in un cono d'ombra proprio in questa legislatura, talvolta avversato e ignorato, quando invece avrebbe dovuto costituire un possibile volano della ripresa economica. Mi riferisco alla realtà portuale di questo Paese. Una realtà che vede mortificata e depressa perfino la propria condizione di vantaggio naturale che gli deriva dall'essere al centro del Mediterraneo e in posizione ottimale per intercettare i traffici che dal *Far-East* scalano i porti europei sulla rotta Suez-Gibilterra. Una realtà che in questi anni si è vista sopravanzare in termini di volumi di traffici da altri porti europei del Mediterraneo, che ha visto aumentare la distanza, ormai siderale, che sempre più ci allontana da quelli del Nord Europa e che si è vista perfino raggiungere dagli scali portuali del Nord-Africa. Una realtà che rischia, se questo Governo non corre rapidamente ai ripari, di subire il colpo di grazia proprio da quello che doveva essere invece l'appuntamento di decollo della nostra economia portuale, ossia la realizzazione delle infrastrutture di valico, Gottardo piuttosto che Sempione o Brennero, e che tra qualche anno, anziché favorire, come era atteso, le rotte dei nostri scali, consentendo alle merci passaggio più agevole oltre le Alpi, costituiranno invece una straordinaria occasione d'ingresso per i porti del Nord-Europa nei confronti del nostro Paese, come in parte avviene già oggi. Nell'attesa disarmante che l'infrastrutturazione dei porti (dal dragaggio dei fondali al banchinamento) e quella necessaria al collegamento tra questi e le principali arterie stradali e ferroviarie diventi priorità riconosciuta finalmente anche da questo Governo, si è assistito a bassezze deplorevoli chi ha cercato di utilizzare il provvedimento milleproroghe come strumento di regolazione dei conti all'interno della compagine di Governo, e tra lo Stato e alcuni territori. Tentativo fortunatamente, e in parte anche misteriosamente, sventato in «zona Cesarini», soltanto pochi minuti prima della presentazione del maxiemendamento. È accaduto infatti che per dare risposta agli impegni assunti da questo stesso Governo (Savona piuttosto che Genova) e per dare soluzione ai problemi determinati dalle attese suscitate e deluse, come nel caso dell'abolizione delle tasse di ancoraggio per i porti di *Transhipment* (vedi Gioia Tauro), scaricando inopinatamente sul sistema i costi della competitività dello scalo, questo Governo intendeva decurtare indiscriminatamente risorse al sistema della portualità, in spregio anche alla legge vigente che consente di redistribuire le risorse, togliendo i finanziamenti ai porti che non sono stati oggettivamente in grado di spenderli. Risorse che peraltro erano state assegnate con specifica legge di finanziamento del settore nel lontano 2002, ma che hanno visto il riparto e l'assegnazione solo due anni più tardi, poi immediatamente congelate dai famosi tetti di spesa, e che soltanto il nostro Governo di centrosinistra ha sbloccato con la finanziaria del 2007. voluti cinque anni per renderle effettivamente disponibile e, dopo soli tre anni, con una norma spregiudicata, si voleva nuovamente requisirle per rimpinguare le casse dell'Erario. Tutto è bene ciò che finisce bene, ed io apprezzo e ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa sorta di miracolo a tempo scaduto, a partire dal Ministero delle infrastrutture per il *forcing* delle ultime ore. Ma mi domando e vi domando: è questa la visione che si ha del Paese? È questa la politica industriale, la politica legata alla logistica dell'Italia? Quella che vede un Governo che, quando non è assente ed ignaro di ciò che si consuma sulla pelle e sopra la testa degli italiani, ci pensa direttamente e per proprio conto a distrarre risorse sugli investimenti che dovrebbero invece costituire il futuro per le nuove generazioni? Questa è l'immagine che si offre agli operatori finanziari ed economici internazionali. Questo, e non altro, è stato invece il senso di emendamenti che sono stati convulsamente presentati da maggioranza ed opposizione, nel disperato tentativo di scongiurare il peggio, costituito da un taglio indiscriminato di circa un miliardo di euro per fare sostanzialmente cassa: emendamenti che alla fine hanno invece avuto successo. In conclusione, siamo - così sembra - alla vigilia dell'esame da parte della 5a Commissione della legge di riforma sulla portualità. Mi permetto al riguardo di rivolgere due accorate richieste, per il valore ed il peso che possono avere. La prima è indirizzata al ministro Tremonti: lo prego di interessarsi, da ora in avanti, con lungimiranza e con l'intelligenza di cui dispone, al settore della portualità, e non con quello spirito avido e rapace che gli è consentito dall'attuale situazione politica ed economica del Paese. La seconda richiesta è rivolta affinché abbia più fiducia nei suoi mezzi. Applichi la legge già in vigore; l'abbiamo fatta noi, quando al suo posto c'era un certo Bersani, credo non a caso. Tolga le risorse ai porti che oggettivamente non li hanno spesi, per proprie deficienze o responsabilità, e faccia ciò che ha in animo di fare senza chiedere indebiti aiuti. Ovviamente, se ne ha la forza, ma anche il coraggio delle proprie responsabilità, cosa che finora non ha sempre dimostrato di avere. *(Applausi Presidente, onorevoli senatori, onorevole rappresentante del Governo, poco fa per i corridoi ricordavo al ministro Vito il diverso atteggiamento di qualche anno fa: quando il buon ministro Chiti veniva a chiedere la fiducia alla Camera, si creavano tumulti in Aula, e lui ne era il protagonista.

tratta, come avevate promesso l'anno scorso o due anni fa, attaccando anche provvedimenti del Governo passato, di un decreto milleproroghe, bensì di una nuova finanziaria con decine e decine di nuovi provvedimenti, provvedimenti, anche sostanziali su alcune materie di cui hanno parlato i colleghi. Credo che - mi rivolgo al Governo - abbiate tradito delle speranze, i risultati sono veramente un disastro per ciò che leggiamo nel maxiemendamento. Il testo iniziale è totalmente stravolto, e ve ne darò degli esempi, soffermandomi soprattutto su alcune materie

di tasse, sia pure complementari per poter ricostruire un territorio, un territorio colpito da una disgrazia? Uccidete l'unità nazionale e l'unico elemento che era rimasto valido per poter tenere unito questo Paese, la solidarietà, che

per altre calamità naturali in cui si è voluto parlare alla comunità nazionale di un Governo efficiente. Non è vero, perché siamo ancora, sia in Abruzzo che nel mio Molise, agli albori della vera e propria ricostruzione.

Sono furbizie che non accettiamo nella maniera più assoluta. Dobbiamo fare qualsiasi cosa per poter tornare indietro.

non avete assolutamente mantenuto. Attendevo in questo provvedimento la risposta alla continuazione della ricostruzione in certe parti del Paese perché, ad esempio, nel Molise siamo al 30 per cento della ricostruzione.

una ricognizione, al di là di come sono stati gestiti certi fondi, che poi appartengono alla vigilanza del Governo passato e di questo Governo? Credo che una ricognizione seria vada fatta perché un diritto alla gente non deve essere assolutamente negato. Avevamo chiesto anche, signor Sottosegretario, di mettere ordine alla confusione sulla restituzione di tributi e contributi: non c'è una norma uguale in tutto il Paese.

diverse che il Governo ha dato negli anni. Bisogna mettere mano alla materia; insediare una commissione per poter dare una risposta che sia una regola. Abbiamo giustamente

e ai familiari delle vittime non è stato assicurato lo stesso trattamento che è stato assicurato alle vittime del gravissimo disastro di Viareggio. Credo che questo Governo non possa fare preferenze in base alle richieste provenienti in quest'Aula. Come pure,

signor rappresentante del Governo, colleghi, desidero rimarcare un aspetto particolare del percorso legislativo di questo provvedimento, che ha visto una cooperazione fra azione del Governo e iniziativa parlamentare anche per la valorizzazione del compito che le Commissioni

In modo specifico, la mia attenzione si riversa sulla Regione Campania e sulla misura contenuta nel decreto-legge in ordine al differimento dei termini dei provvedimenti concernenti le demolizioni delle costruzioni abusive. in questi giorni si è acceso anche un forte dibattito nel Paese e sulla stampa, con dichiarazioni talvolta anche forti nei toni, ma che - a mio avviso - merita un'attenzione particolare e soprattutto un approfondimento in termini concreti

una inazione che ha riguardato innanzitutto i livelli locali, e quindi le amministrazioni locali, le Regioni e le Province nelle rispettive competenze in materia di potestà pianificatoria. Ha riguardato però anche le altre autorità preposte ai controlli, perché altrimenti mai si sarebbe potuto sviluppare un fenomeno di tali dimensioni. Questa vicenda ci insegna anche un'altra cosa, sulla quale è opportuno fare chiarezza: la demagogia, le strumentalizzazioni e soprattutto le valutazioni ancorate ancorate ad una visione dogmatica, alla prova dei fatti, non reggono. Tutto questo nasce da una particolare vicenda della produzione normativa della Regione Campania che, con una dichiarazione molto opinabile sul piano dei contenuti, nel 2004, attraverso un semplice atto deliberativo, ossia una delibera di Giunta regionale, dichiarò inapplicabile l'istituto del condono nella Regione stessa. Si tratta di un provvedimento francamente

La Regione reiterò, questa volta attraverso un intervento legislativo, una definizione di criteri, di principi e di parametri applicativi dell'istituto della sanatoria, altrettanto stringenti e forse per certi versi ancora di più. Anche in questo caso - peraltro l'intervento avveniva fuori termine - il Governo del tempo si rivolse alla Corte costituzionale, la quale con un'ulteriore pronuncia, per l'esattezza la n. 49 del 2006, ribadì l'illegittimità di questo intervento normativo. Dopodiché, ovviamente i giudizi penali, nel frattempo promossi e attivati, sono andati avanti, non essendo stato possibile per i cittadini di quella Regione l'utilizzo dell'istituto della sanatoria che una legge dello Stato garantiva a tutti i cittadini della Repubblica. Conseguentemente, oggi siamo nella fase dell'esecuzione. Molto opportunamente in questa misura si prevede che la Regione Campania ridefinisca il sistema vincolistico attraverso una ridefinizione dei piani paesaggistici. Dobbiamo ricordare che ancora una volta, rispetto ai piani vigenti, si sconta una inerzia dell'amministrazione. Infatti, oltre dieci anni fa, da parte del Ministero dei beni culturali ci fu il commissariamento nella redazione di questi strumenti di pianificazione, non sempre si è tenuto conto dell'effettiva consistenza dello stato dei luoghi e soprattutto del grado di pregio ambientale che determinate aree rivestono. Pertanto, ancorare oggi il differimento delle esecuzioni ad un tempo ragionevole - dieci mesi - che permetterà alla Regione Campania di ridefinire i piani paesaggistici, significa cominciare finalmente a riportare ordine e legalità in un settore dove il disordine, la confusione e la sovrapposizione di norme confuse e spesso - come poi la Corte costituzionale ha potuto sancire - assolutamente illegittime hanno concorso non poco a generare un fenomeno di dette dimensioni, che ci auguriamo vivamente e sentitamente non abbia più a ripetersi nella nostra Regione. Soltanto per questo, ovviamente rispetto alle tante altre misure poste nel provvedimento a sostegno

Signora Presidente, onorevoli colleghi, affronterò soltanto un punto di questo provvedimento, sul quale è stata posta la fiducia, e intendo farlo perché è stata commessa un'azione ingiusta, nonostante le promesse solenni fatte poco tempo fa. Mi riferisco alla materia della media conciliazione. L'avvocatura ha salutato favorevolmente l'introduzione di questo nuovo istituto, ponendo però due questioni di fondo: la mediazione-conciliazione può essere un modo deflattivo del contenzioso civile, ma è necessario che venga garantita la professionalità del mediatore e del conciliatore, nonché l'assistenza tecnica delle parti. Poi è all'evidenza da escludere una obbligatorietà La legge delega, infatti, non prevedeva l'obbligatorietà. Il provvedimento del Governo invece inserisce l'obbligatorietà, che si traduce in qualcosa di estremamente semplice: un cittadino con le sue pene si reca da un avvocato, gli racconta i suoi problemi, gli mostra le sue carte, chiede assistenza per la tutela di un diritto che ritenga violato. L'avvocato lo ascolta e poi gli dice: «In questo momento e da questo momento la mia attività si è esaurita perché la sua controversia dovrà essere risolta da un mediatore. Chi esso sia non si sa, ma da un mediatore. potrà anche non accettare la soluzione, però obbligatoriamente deve ricorrere al mediatore. Le viene imposto per legge, e se non fa il ricorso al mediatore lei non potrà mai chiedere la tutela di un proprio diritto ad un giudice». Criticando questi due aspetti della soluzione proposta dal Governo, il Ministro della giustizia, al Congresso nazionale forense dello scorso novembre, tenutosi a Genova, assunse il formale impegno di ridiscutere questi due punti critici del provvedimento. Assunse un formale impegno, capendo che erano temi delicati da affrontare e comprendendo che dietro ogni questione c'è un diritto e dietro un diritto ci sono le interpretazioni, le norme, i codici. Non esiste una giustizia che amministri un diritto senza forme, senza codici, senza assistenza tecnica. Diversamente, avremmo i capi tribù che un giorno al mese raccolgono il popolo al centro del paese per amministrare giustizia e dispensare diritti e doveri. invece, dopo le promesse, siamo arrivati alla soluzione per cui l'istituto, con le caratteristiche di obbligatorietà e di non assistenza tecnica, entra in vigore, pur accantonandosi per il momento che esso possa essere applicato a determinate fattispecie di contenzioso, in materia condominiale e di responsabilità della circolazione dei veicoli e dei natanti. Ma l'istituto, così com'è, entra in vigore, e invece bisognava discutere proprio dei suoi contenuti, e in modo particolare del requisito dell'obbligatorietà della giustizia alternativa, di questa giustizia che viene privatizzata.

Ma questa non è amministrazione del diritto: questa è la privatizzazione della giustizia e la rottamazione del processo civile. Non è una riforma: è tornare ad una giustizia tribale! Per questo, noi

si era posta una condizione, con l'approvazione di un emendamento che prevedeva uno slittamento di ulteriori 12 mesi, perché nel frattempo si potesse discutere di questi profili delicati.

perché non può parlarsi di riforma quando un cittadino, che chiede la tutela di un proprio diritto,

- cioè alla vendita dei diritti in mano a chi il diritto non conosce, a chi non deve applicare né codici, né norme, né giurisprudenza, né procedure. Tutto liberalizzato! L'Italia, culla del diritto, rinnega il diritto, perché ritiene la forma del processo un orpello inutile del quale si può fare a meno. Questa è un'espressione di disprezzo profondo verso la nostra tradizione giuridica, e giustamente

Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, un nostro emendamento al decreto in discussione chiede di mantenere le attuali graduatorie provinciali degli insegnanti precari fino al 31 agosto 2012.

La nostra richiesta, da realizzarsi ovviamente «fatti salvi gli adempimenti conseguenti alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4-*ter* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167», ha le stesse motivazioni. Non sappiamo ancora quanti insegnanti grazie all'ultima sentenza della Consulta, potranno inserirsi "a scavalco" nelle graduatorie. È certo però che diversi docenti, non solo del Centro-Nord, che negli ultimi anni, pur precari, hanno lavorato in maniera continuativa, perderanno il posto (cosa che a una parte della sinistra pare proprio non interessare). Questo in conseguenza di punteggi abnormi (a volte più che doppi, e non capiamo come mai a chi straparla di merito non venga qualche dubbio su certi numeri, che danneggiano prima di tutto le persone serie del Sud) maturati in alcune aree del Paese da molti di coloro ai quali è stato consentito di iscriversi come riserva nelle graduatorie di altre Province. Ora viene imposto che questi docenti si possano riposizionare su una graduatoria diversa da quella originaria, inserendosi a pettine, cioè in base al punteggio, stravolgendo le liste e facendo saltare quello che chi era già presente in graduatoria considerava ormai un diritto acquisito. Un diritto reale, stando alle parole di Fioroni nel 2007, ma che rischiava di svanire del tutto senza l'intervento dell'emendamento che abbiamo inserito nel provvedimento in discussione che limita le conseguenze della sentenza della Consulta a coloro che hanno presentato ricorso. Ora, se davvero, come dice la Corte costituzionale, si vuole valorizzare il merito, va riformato con la massima urgenza il meccanismo di reclutamento degli insegnanti. Abbiamo già consegnato al ministro Gelmini una proposta articolata, sulla quale le principali forze sindacali, CGIL esclusa, hanno manifestato disponibilità. Proponiamo un meccanismo su base regionale, ma non ci sono fili spinati. Il progetto, che non ha nulla di discriminatorio nei confronti di nessuno, come invece vorrebbe dare ad intendere qualcuno, è in linea con la Costituzione, la legge nazionale e la normativa europea. Per assegnare il punteggio di base ai candidati non si farà più riferimento, se non in misura ridotta, alla valutazione acquisita sul proprio territorio. Si dovrà scegliere una e una sola Regione nella quale eleggere il proprio domicilio professionale e sottoporsi a quello che abbiamo chiamato test di preparazione con cui si verificherà la attitudine all'insegnamento e l'effettivo livello di preparazione dei candidati nelle singole materie. Il tutto - questo è il punto fondamentale - nella Regione di arrivo, a parità di condizioni con i candidati del posto. Chi è stato valutato in maniera troppo generosa in altre realtà, non potrà più scavalcare chi effettivamente merita, sia che venga dal Nord, sia che venga dal Centro, sia che venga dal Sud. Signora Presidente, interverrò su due specifiche questioni trattate nell'ambito delle due Commissioni riunite e riproposte nel maxiemendamento del Governo. La prima questione attiene ad un regalo che questo Governo ed in particolare il Ministro dell'agricoltura intendono fare ad alcuni ricchi miliardari veneti, possessori di valli da pesca nella laguna di Venezia. Da alcuni decenni assistiamo a processi penali, civili, amministrativi e contabili che riguardano l'abusivo impossessamento di spazi demaniali della laguna da parte di privati. Fino dall'epoca della Serenissima Repubblica di Venezia, detti spazi erano ritenuti di proprietà pubblica, proprietà ribadita anche all'epoca delle successive invasioni francesi e austro-ungarica, nonché dallo Stato sabaudo ed infine dalla Repubblica italiana. La magistratura repubblicana fino ad ora ha, per lo più, confermato tale natura pubblica di acque e spazi lagunari. In Commissione agricoltura del Senato sono pendenti e in elaborazione due disegni di legge al fine di regolamentare la materia a favore soprattutto di piccoli imprenditori che coltivano per davvero le terre bonificate e che noi del PD intendiamo davvero tutelare. E su questi disegni di legge, la Commissione giustizia del Senato, preventivamente e all'unanimità, con il relatore Mazzatorta, capogruppo in Commissione della Lega Nord, richiamando il disegno di legge n. 1239, di cui il sottoscritto ha scritto nel proprio parere alla Commissione agricoltura che «le valli da pesca della laguna di Venezia e di Marano devono essere considerate come appartenenti *ab origine* al bacino demaniale marittimo delle lagune stesse». Ora, che cosa fa il Governo, invece di tutelare il patrimonio pubblico? Dopo aver sottratto, con un improvvido tratto di penna, il Canal Grande ai veneziani, questo Governo e questa maggioranza tentano di sottrarre al demanio pubblico le valli da pesca abusivamente occupate da pochi privilegiati, cercando di anticipare l'attuazione dei decreti sul cosiddetto federalismo demaniale. Ma lo fanno, peraltro, con un emendamento che sarebbe probabilmente inammissibile perché *extra materiam*, con un *escamotage* giuridico che, purtroppo per loro, essendo tecnicamente scritto male, darà origine ancora una volta a contestazioni e processi. Alla faccia del cosiddetto federalismo, alla faccia della tutela dei beni pubblici, ancora una volta nell'ottica di favorire pochi privilegiati, ai danni dei cittadini e delle amministrazioni territoriali! La seconda questione attiene alla cosiddetta mediazione-conciliazione, istituto giuridico richiesto da tempo, soprattutto in vista di un consistente effetto deflattivo sul numero dei processi civili.

il proprio parere favorevole alla necessità di una congrua proroga, «in considerazione dell'ampio consenso intorno alla necessità di una revisione di questa materia prima della sua definitiva entrata in vigore».

tanto che ora ci troviamo di fronte ad un emendamento del Governo, all'interno del maxiemendamento, che viene decisamente contestato in particolare da tutte le organizzazioni e dagli organismi forensi, oltre che dagli altri operatori della giustizia. Probabilmente, al Governo e al suo Ministro della giustizia interessa non tanto far funzionare la macchina della giustizia civile, quanto piuttosto poter piantare una piccola bandierina propagandistica. Che poi l'istituto della mediazione-conciliazione funzioni o meno, che le strutture non esistano, che le garanzie non ci siano, che il personale non esista, che la formazione non esista, al Ministro non interessa. E, fatto ancor più grave, sembra che al Ministro della giustizia non interessino nemmeno il rispetto della Costituzione e la tutela dei diritti della difesa, gravemente menomati da questo decreto, come denunciato chiaramente anche dagli organismi forensi, oltre che dai senatori della Commissione giustizia, i quali tutti - maggioranza e opposizione

Evidentemente, Governo e Ministro della giustizia non sono interessati. Prendiamo atto che privilegiano altre logiche, anche scontrandosi con il Parlamento, imponendo per di più ripetuti voti di fiducia. Confidiamo che ciò succeda ancora per poco e che questo Governo tolga le tende e se ne vada. *(Applausi

Governo e Parlamento utilizzano una legge veicolo nella quale trovare una compiuta risposta a precisi e specifici problemi del Paese che, difficilmente, per la loro particolarità, potrebbero avere altra sede nei provvedimenti parlamentari.

questione di fiducia, come se l'esistenza di un provvedimento capace di offrire soluzioni ad una miriade di questioni sia di per sé un difetto. Da parte di chi cerca comunque ragioni per opporsi ad ogni iniziativa del Governo e della maggioranza prevale, quindi, l'argomento di una contestazione formale sulla tecnica legislativa. Presidente, che sostanzialmente e concretamente nel decreto che oggi approviamo rinnovando la fiducia al Governo trovino risposta e soluzione molti bisogni, trovino risposta e soluzione molti bisogni, molti problemi di questa Italia, quelli di cui tutti dicono di voler parlare, che sono però relegati ai margini del dibattito politico e dell'attenzione dei *mass-media* rispetto ad altri argomenti che, ahimè, perfino oggi si sono voluti tirare dentro ad un dibattito parlamentare che con essi non ha proprio nulla a che fare. Altri colleghi hanno parlato e parleranno delle molte questioni sulle quali il provvedimento in esame dà compiute risposte, del ripristino di una quota sostanziosa del finanziamento del cosiddetto 5 per mille a fondazioni ed associazioni meritorie. Altri colleghi parleranno del finanziamento per i sistemi portuali e dei soldi per la cultura. Desidero come senatore eletto in Liguria esprimere la mia e nostra soddisfazione, unitamente ai colleghi Bornacin e Boscetto, per il finanziamento di 90 milioni di euro per i gravi danni connessi agli eventi alluvionali che hanno colpito nei mesi scorsi la nostra Regione. La Liguria, piccola Regione con molti problemi, prima di questo provvedimento non aveva trovato uno stanziamento adeguato per le infrastrutture, i beni pubblici e privati gravemente compromessi da eventi alluvionali. Eppure ancora oggi nella mia provincia, dopo quasi due mesi dall'evento, c'è una importante strada che è totalmente interrotta per una frana ed intere comunità sono condannate a percorrere ore di automobile per raggiungere scuole e posti di lavoro accessibili attraverso la strada interrotta in soli pochi minuti. In cittadine come Varazze, nel Ponente Genovese e nello Spezzino, le risorse assegnate fino ad oggi non sono bastate neppure per eliminare i detriti degli smottamenti e per ripristinare la sicurezza idraulica dei torrenti esondati. Arrivano i soldi per risolvere questi gravi problemi e molti liguri ritrovano, grazie a questo provvedimento, alla maggioranza ed al Governo che lo sostengono, una speranza per il loro futuro. Un mese fa, con gli altri colleghi parlamentari del PdL eletti in Liguria, abbiamo scritto una lettera al Presidente del Consiglio, con contenuti e toni anche risoluti per richiedere un suo personale impegno per garantire una copertura finanziaria alle richieste di stanziamento. Con il parere favorevole che il Governo ha espresso sull'emendamento votato in Commissione ed oggi riproposto nel maxiemendamento governativo, è giunta la risposta che ci attendevamo. Per questo dobbiamo ringraziare il Governo ed i relatori. Per la convinzione sulla necessità di rinnovare la fiducia a questo Governo esprimerò ed esprimeremo la nostra fiducia, e, sia chiaro, lo avremmo fatto comunque per continuare ad onorare quell'impegno che abbiamo personalmente assunto con i nostri elettori; ma credo lo faremo anche con la grande soddisfazione di aver dato una risposta ad un problema grave delle comunità che che ci hanno eletti. Ringraziamo quindi tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato, frutto anche di un gioco di squadra, indipendentemente dagli schieramenti politici, dal presidente della Regione Burlando, ai colleghi senatori liguri eletti anche in altri schieramenti, che con noi hanno sollecitato e proposto il finanziamento. Sta di fatto però che oggi, una maggioranza vota anche per le risorse delle alluvioni e un'opposizione vota contro e, grazie al nostro voto, al voto della maggioranza, si allungherà con questo provvedimento la lista delle piccole e grandi cose positive che in questi quasi tre anni sono state realizzate. Siamo convinti che questa soddisfazione nel contribuire a fare cose positive sia ciò che conta, ciò che gli italiani si aspettano da noi e ciò che nobilita la funzione della politica, ciò per cui dobbiamo proseguire nel cammino del Governo del Paese.